Onorevoli senatori, ricorre oggi il centesimo anniversario della nascita della nostra illustre collega, la professoressa Rita Levi-Montalcini. Per ragioni strettamente personali ella non ha potuto accogliere il mio invito ad essere oggi presente tra noi. Le consegnerò pertanto, nei prossimi giorni, una medaglia celebrativa di questa bella ricorrenza. Sarà questo un doveroso segno di omaggio e di augurio da parte dell'istituzione che la accolse tra i suoi membri per decisione del capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, in virtù degli altissimi meriti in campo scientifico e sociale con i quali ha saputo illustrare ed onorare l'Italia. Il suo contributo scientifico, che ha fatto di lei una figura nota ed apprezzata in tutto il mondo e che le ha guadagnato l'altissimo onore di essere insignita del premio Nobel per la medicina nel 1986 (diciassettesimo cittadino italiano a ricevere tale importante riconoscimento), non esaurisce però la multiforme ricchezza di questa straordinaria figura di donna e di scienziata. Rita Levi-Montalcini è infatti per tutti noi, prima ancora che una grande scienziata, una preziosa testimone di quello spirito di intelligenza, di tenacia, di umiltà e di responsabilità sociale che si rivela, in ogni ambito dell'agire umano, lo strumento indispensabile per superare le difficoltà e conseguire i risultati più difficili e insperati. Fu grazie a questo spirito tenace e coraggioso che una giovane e brillante studiosa seppe reagire all'infamia delle leggi razziali rifiutando di cadere nell'amarezza e nel distacco e trasformando quella difficile situazione in una opportunità per intraprendere, seppure in circostanze fortunose e precarie, nuove esperienze di ricerca al di fuori dei circuiti accademici. Negli anni successivi, al termine di un fecondo periodo di ricerca negli Stati Uniti e in Sud America, quella stessa studiosa diede una grande prova di amore per il suo Paese, nonché di consapevolezza della responsabilità sociale dell'uomo di scienza, decidendo di tornare a casa e trasmettere alla nostra comunità scientifica quanto aveva saputo realizzare, contribuendo così in maniera determinante a impiantare e a sviluppare qui in Italia strutture di ricerca che sono oggi all'avanguardia nel mondo. Con lo stesso spirito di generosa apertura alla condivisione del proprio sapere e delle proprie conquiste, ella alimenta ancora oggi, accanto al lavoro scientifico, una vigorosa attività editoriale di divulgazione del metodo e delle ragioni della scienza nei confronti del grande pubblico. A questa preziosa opera di divulgazione si affianca l'azione quotidiana della Fondazione Levi-Montalcini - nel cui logo significativamente campeggia il motto «Il futuro ai giovani» - orientata, fra l'altro, all'assistenza delle giovani generazioni nella scelta del percorso di studio e di lavoro attraverso una rete di centri di orientamento, nonché alla valorizzazione del contributo femminile al progresso della società, in particolare nei Paesi di via di sviluppo, attraverso la formazione culturale e professionale delle giovani donne. Tutte queste iniziative si alimentano nella consapevolezza costante che, come ha dichiarato la nostra illustre collega, fare scienza non è altro che esercitare il desiderio di aiutare gli altri. E allora è con grande affetto, certo di interpretare il sentimento unanime di tutta l'Assemblea, che rinnovo a Rita Levi-Montalcini l'omaggio e l'augurio del Senato della Repubblica, che si onora oggi di annoverarla tra i suoi membri.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei giorni scorsi la Corte suprema dell'Iran ha concesso di sospendere per alcuni giorni l'esecuzione di una sentenza di condanna a morte nei confronti di una cittadina iraniana, Delara Darabi, che all'epoca del reato che le è stato attribuito era minorenne. Questa ragazza, che aveva 17 anni nel settembre del 2003, insieme al suo fidanzato,

la ragazza. Questa si fece carico di attribuirsi la responsabilità di quell'omicidio, convinta che con tale affermazione avrebbe salvato la vita al suo fidanzato. Ci sono prove anche di questo, legate al fatto che, secondo la perizia, l'omicidio non poteva essere stato compiuto che da una persona destrorsa, mentre la ragazza è mancina. È iniziata, da quel momento una vicenda giudiziaria lunga, complessa, delicata e difficile.

Il ragazzo è stato condannato a 10 anni di carcere e sono stati entrambi condannati a essere frustati per relazione illecita. La sentenza avrebbe dovuto essere eseguita questo lunedì. Vi è stata una mobilitazione, assolutamente priva di colore politico, in moltissimi Paesi del mondo occidentale, e non solo, perché quella sentenza non venisse eseguita. Voglio ricordare, in particolare, che si tratta di una condanna a morte nei confronti di una minorenne

norma del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia che vieta di eseguire condanne a morte nei confronti dei minori. Noi abbiamo seguito con molta attenzione quanto sta accadendo in queste settimane nell'ambito delle relazioni tra il mondo occidentale e l'Iran. Siamo convinti che proseguendo sulla strada intrapresa del dialogo, nonostante le preoccupazioni di questi giorni per alcune inaccettabili affermazioni del presidente Ahmadinejad,

possa intervenire presso il Governo italiano e il Ministero degli affari esteri al fine di esercitare ogni legittima pressione nei confronti dell'Iran perché la sentenza non sia eseguita.

La legge islamica in vigore in Iran prevede la piena imputabilità dei cittadini minorenni: dall'età di 9 anni fino ai 13, se di sesso femminile, e dai 15 anni se di sesso maschile. In Iran sono state eseguite, nel 2008 e nel 2009, già nove condanne a morte di

della giovane iraniana Delara Darabi per un delitto commesso all'età di 17 anni. Bisogna inoltre tener conto del fatto che per Delara Darabi sono già stati esperiti tutti i gradi di giudizio e che quindi ormai la condanna è è inappellabile. L'esecuzione di un condannato che fosse minorenne all'epoca del reato è proibita dal diritto internazionale, così come dichiarato nel Patto internazionale sui diritti civili e politici

confronti delle autorità politiche iraniane affinché venga commutata la condanna a morte di Delara Darabi, a prescindere dall'ottenimento del perdono dei familiari della vittima, come previsto dalle norme di diritto internazionale a tutela dei minori.

avvalersi delle professionalità che si sono già formate. In particolare, vi è l'esigenza di assumere, in questo contingente, i volontari in ferma breve delle Forze armate già vincitori di concorso, che sarebbero stati esclusi dal bando che

me, vantino un diritto quesito ad essere assunti dalla pubblica amministrazione, proprio perché la formazione professionale di queste forze è straordinariamente necessaria per il contrasto di illeciti

Il senatore Saltamartini lo sa bene.

Dichiaro chiusa la votazione. **Il Senato non approva.**

Dichiaro chiusa la votazione. **Il Senato non approva.**

degli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa. Se si eliminasse l'ultimo periodo prima del dispositivo, il parere sarebbe favorevole.

precisate come al di là da venire. Visto che si è voluta inserire una norma a tutela dei lavoratori delle forze di polizia e delle Forze armate, e in particolare per i casi di infortunio sul lavoro e di malattie professionali, riteniamo che tutti i lavoratori siano uguali e che quindi per tutti i lavoratori debbano valere le medesime norme, anche nel caso della situazione prevista dal

agiscono anche in scenari esteri, che possono essere colpite da patologie quali quella dell'uranio impoverito, chiediamo che vengano applicate le norme più favorevoli.

il termine a partire dal quale i gestori telefonici devono rendere disponibili alla polizia e all'autorità giudiziaria i dati di traffico telefonico relativi alle chiamate senza risposta.

da rete mobile o da rete fissa, la condizione di illegittimità comunitaria in cui versa la nostra normativa sul punto, dal momento che le norme sulla fornitura da parte dei gestori dei dati relativi al traffico telefonico, anche se relativi alle chiamate senza risposta, avrebbero dovuto essere applicate dal gennaio del 2008, data dalla quale è ormai passato un anno e mezzo. Si consideri, inoltre, che tale differimento nel tempo della fornitura di tali dati da parte dei gestori telefonici rischia di pregiudicare gravemente importanti indagini giudiziarie, a discapito ovviamente della sicurezza pubblica. Per mia memoria, ma anche per la memoria di tutti, ricordo che gli attentati terroristici di Londra e di Madrid sono stati causati dall'innesco di esplosivi reso possibile da una chiamata senza risposta. Con questa norma si allungano ancora i tempi per poter intervenire nei casi di chiamate di questo genere, rendendo maggiormente

direttiva Frattini, al fine di non pregiudicare le indagini che potrebbero invece avvalersi di tali dati. L'emendamento 12-*ter*.4 mira a sopprimere una norma introdotta dal decreto milleproroghe, gravemente lesiva della *privacy* dei cittadini, nella misura in cui liberalizza le chiamate di disturbo a tutto vantaggio dell'industria del settore e a tutto svantaggio della riservatezza individuale. finestra"). Colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti della scuola secondaria di primo grado «Ascanio Grandi» di Lecce. Diamo il benvenuto a loro e ai loro insegnanti.

dei dati che, com'è noto, è di 24 mesi per i dati di traffico telefonico, 12 mesi per i dati di traffico telematico e 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta, senza distinzioni in base al tipo di reato.

premesso che il comma 2 dell'articolo 12*-ter* del provvedimento in esame stabilisce che, per quanto riguarda le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009. Il comma 3 stabilisce invece che, per quanto concerne le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010; impegna il Governo a vigilare, monitorare e valutare ogni eventuale verifica e misura in relazione all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 12-*ter*.

e la formazione di personale delle forze di polizia provenienti dalle forze armate, impegna il Governo, salvaguardando in ogni caso i diritti quesiti dei candidati di concorsi già banditi o in via di emanazione, a valutare l'assunzione dei volontari in ferma breve risultati idonei ma non vincitori di concorso.

rispetto al quale diamo atto al ministro Carfagna di aver svolto un buon lavoro, anche se i tempi ristretti concessi al Senato per l'esame di questo decreto non hanno consentito di migliorare la nuova figura di reato che è stata introdotta riguardante

norma. Apprezzo altresì la circostanza che la maggioranza e il Governo hanno fatto un passo indietro su due disposizioni contenute in questo decreto che più che servire al contrasto dell'immigrazione clandestina servivano a soddisfare alcune esigenze politiche interne alla maggioranza. che estendeva in maniera indiscriminata il tempo di permanenza nei centri di identificazione, senza che ciò fosse agganciato ad una rivisitazione della normativa che riguarda più complessivamente il contrasto all'immigrazione clandestina, ed alla norma che riguarda l'istituzione delle cosiddette ronde, che poco servono al sistema della sicurezza, anche perché il mondo del volontariato è già impegnato a a sostenere le attività istituzionali dei Comuni: lo fa nel settore della protezione civile, dell'assistenza e della solidarietà sociale ed, anche, ancorché in una misura più ristretta, nell'ambito di ciò che attiene ai compiti di sicurezza, propri della polizia amministrativa locale.

rappresentano però un passo avanti e positivo nel contrasto ad alcune forme di reato e, quindi, ci mettono nella condizione di votare a favore. Aspettiamo con ansia che il Governo sottoponga all'esame del Parlamento una proposta reale e complessiva sui temi dell'immigrazione a partire, ad esempio, dal recepimento della a partire, ad esempio, dal recepimento della direttiva rimpatri, pubblicata nel dicembre 2008 - ed in quella sede si potrà aprire un confronto sui temi di estrema attualità, visto il moltiplicarsi degli sbarchi e degli ingressi illegali e ci metta anche nella condizione di esaminare con attenzione un'attenta rivisitazione della legge Bossi-Fini, rivisitazione auspicata peraltro anche da uno dei padri putativi di questa legge, cioè l'attuale Presidente della Camera. Per queste ragioni, signora Presidente, togliamo il disturbo e votiamo a favore di questo provvedimento. *(IdV)*. Signora Presidente, come già detto nel corso della discussione generale, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha ritenuto

e condizionato questo provvedimento, che è già operativo sul territorio nazionale.

Contesto radicalmente questa affermazione, perché se il Governo e la maggioranza avessero avuto effettivamente tale sensibilità, questa norma sarebbe già parte del nostro sistema, sin dal luglio dello scorso anno. Anzi, sarebbe stata una norma scritta meglio, perché su di essa dovremo reintervenire per modificarla, quanto è stata formulata male rispetto alle previsioni contenute nei testi dei disegni di legge dell'opposizione, che riprendevano disegni di legge del Governo della scorsa legislatura. Se il Governo e la maggioranza avessero veramente avuto a cuore i problemi dei cittadini voluto manifestare sensibilità verso una forma di criminalità sicuramente allarmante, prodromica ad atti di violenza spesso diffusi, avrebbero approvato quella norma quando venne presentata nel luglio del 2008 e si sarebbero evitati degli omicidi. Quindi, se c'è qualcosa che rimproveriamo al Governo ed alla maggioranza è la mancanza di sensibilità su un tema caldo. ragione tutto ciò che è avvenuto dal luglio 2008 fino al febbraio 2009 in mancanza di questa norma è colpa vostra, è a voi ascrivibile, altro che sensibilità. Si tratta invece di un'iniziativa che si deve ascrivere alla tendenza ormai ampiamente diffusa e conclamata del Governo non volere consentire che i disegni di legge e le proposte di iniziativa parlamentare possano vedere la luce in un'Aula parlamentare, attraverso un percorso rispettoso delle prerogative del Parlamento. Il Governo si appropria della materia proposta dai parlamentari, se ne appropria spesso male e la propone sotto forma di decreto. Noi denunziamo quindi tale espropriazione delle prerogative parlamentari, sapendo anche che probabilmente i nostri Regolamenti consentono che si possa violentare l'iniziativa del Parlamento. Anche se ci fosse una maggiore attenzione nell'applicazione dei Regolamenti, ed in modo particolare dell'articolo 51 alcuni problemi li potremmo gestire diversamente. L'articolo 51 valorizza il lavoro del Parlamento e l'iniziativa dei parlamentari, dando facoltà al Governo, qualora intenda presentare un disegno di legge sulla medesima materia, di chiedere un rinvio di un mese della trattazione. Invece attualmente i nostri disegni di legge, già pronti per il voto in Aula a seguito dell'esame in Commissione, rimangono parcheggiati, dal mese di novembre dello scorso anno, in quanto il Governo ha annunciato di voler intervenire sulla medesima materia, ed ancora, a distanza di circa sei mesi, non lo ha fatto. E questo si ripete in molte circostanze. Denunziamo quindi ciò che è avvenuto attraverso questo provvedimento, che non è ascrivibile a nessuna sensibilità ma esclusivamente alla voglia di inscrivere l'intervento tra le iniziative di natura mediatica del Governo, che deve comunque presentarsi agli italiani

aumentare quelle forme di discredito e di critica che da parte dell'opinione pubblica investono le istituzioni alte.

Signora Presidente del Senato, signori senatori, signori del Governo, il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, dall'inizio del suo *iter* parlamentare è stato trasformato e, per così dire, ha cambiato pelle. Era stato presentato con molta enfasi dal Governo e da questa maggioranza come risolutivo nella lotta contro la criminalità e l'immigrazione clandestina. Era stato fatto passare presso l'opinione pubblica questo messaggio con la precisazione nella proposta di due norme manifesto sulle cosiddette ronde e sui centri di identificazione ed espulsione, norme propagandistiche - soltanto propagandistiche - inutili in concreto e per di più, almeno quella sui centri di identificazione ed espulsione, in aperto contrasto con la normativa europea. A quest'ultimo proposito va decisamente contestata l'interpretazione della normativa europea fornita anche in quest'Aula ieri, in particolare dai rappresentanti della Lega Nord, il cui ordine del giorno è stato accolto dal Governo. Non è assolutamente vero che la norma sui CIE, prevista all'articolo 5 del decreto-legge, cassato alla Camera dei deputati dalla stessa maggioranza, corrisponde alle direttive europee in quanto assolutamente diversi sono i presupposti giuridici. Infatti, il termine massimo di detenzione nei CIE, fissato in 18 mesi dalla direttiva comunitaria in materia di ingressi invocata dalla Lega, vale per i casi di resistenza all'identificazione ma non anche per i casi di difficoltà nell'accertamento dovuti magari a negligenze o inefficienze di organi amministrativi italiani o stranieri. Non è accettabile una detenzione amministrativa di 6 o peggio di 18 mesi sulla base di un requisito, quale il ritardo nell'acquisizione di documenti, del tutto estraneo al comportamento del singolo soggetto. Tra l'altro, è la stessa commissione De Mistura a dimostrare e a dichiarare che i tempi tecnici per l'identificazione dello straniero non superano i 60 giorni. Come si fa a giustificare una reclusione per mesi e mesi nei confronti di chi non abbia commesso nessun delitto, sulla base, per di più, di circostanze estranee alla sua condotta e a seguito di una procedura che appare priva dei requisiti di garanzia richiesti dalla direttiva? Ricordiamoci che in altri Stati europei, come ad esempio la Germania e in tutto il Regno Unito, la detenzione per più di 15 giorni è subordinata alla dimostrazione in giudizio da parte dell'autorità amministrativa di aver diligentemente compiuto le operazioni necessarie all'identificazione, non potendosi addossare allo straniero le conseguenze di negligenze o inefficienze dei vari Stati e polizie. Signori del Governo, se la settimana prossima per davvero dovranno essere rilasciati cento o mille stranieri, la colpa non sarà della mancanza di leggi adeguate o dell'opposizione: la colpa sarà tutta vostra e deriverà dal fallimento della politica di sicurezza in questo anno del vostro inefficiente Governo e nei cinque anni del precedente Governo Berlusconi, che ha saputo partorire soltanto una legge, la cosiddetta criminogena e causa, a sua volta, di illegalità irrisolte e forse irrisolvibili. Per buona sorte, ci ha già pensato la Camera dei deputati a cassare queste due indecorose norme su i CIE e sulle ronde. Questo è il motivo principale per cui del decreto‑legge al nostro esame si può dire ora: c'era una volta. Nell'altro ramo del Parlamento il Partito Democratico ha votato a favore delle rimanenti norme del decreto‑legge perché formulate in ordine a gravi e delicati fatti di criminalità che, ripetutamente, con pesante costanza colpiscono donne, bambini e persone deboli. Nessuno può nascondere che le violenze sessuali sulle donne e sui minori, così come gli atti persecutori, siano diventate una piaga insopportabile ed inaccettabile per il nostro Paese, come per ogni Paese civile. È evidente, quindi, la necessitàdi intervenire in materia con una nuova e specifica regolamentazione dal punto di vista sia del diritto sostanziale che di quello processuale. Il Partito Democratico si era già fatto carico di tali esigenze predisponendo e presentando, anche in Senato, specifici disegni di legge sulla violenza sessuale di gruppo e monosoggettiva, sui maltrattamenti in famiglia, sulla violenza ai danni di minori e sul cosiddetto *stalking*. Ora abbiamo assistito ad un'opera un po' arlecchinesca da parte del Governo che, in un unico decreto‑legge, aveva inserito norme diverse tra loro, con finalità molto diverse, e con beni giuridici da tutelare e strutture di reato un po' raffazzonate. Governo l'importante non era e non è risolvere i problemi quanto piuttosto far credere all'opinione pubblica di avere in mano quasi una bacchetta magica.

Sgombrato allora il campo dalle due citate norme su ronde ed espulsioni, grazie soprattutto - lo ricordo e lo sottolineo - a spaccature nella maggioranza analogamente a quanto era successo sulla stessa materia in questa Aula alcune settimane fa discutendo del disegno di legge n. 733, va segnalato che l'odierno provvedimento legislativo tende positivamente a rafforzare gli strumenti sostanziali e processuali per contrastare ogni forma di aggressione sessuale notoriamente realizzata nei confronti di soggetti deboli. I tempi ristretti di un decreto-legge e la tecnica legislativa da Arlecchino del Governo hanno, peraltro, condotto alla redazione di un testo che, se accettabile nelle sue linee generali, lo è molto meno nei particolari e in quella necessaria determinatezza e precisione delle fattispecie degli istituti che sarebbero richiesti. Riteniamo che l'approvazione oggi di questo decreto-legge sia soltanto un primo passo a tutela delle donne e dei minori, un primo passo importante, ma ancora e certamente insufficiente. In questo senso va colta positivamente la disponibilità del relatore, anche se non abbiamo sentito nello stesso senso la disponibilità del Ministro intervenuto ieri in questa Aula. In questo decreto-legge la caratteristica predominante è quella dei chiaroscuri. Se va sicuramente ben accolta la norma che autorizza in sostanza l'immissione in servizio permanente di nuovo personale, in particolare nell'Arma dei carabinieri, rimane incomprensibile però l'indisponibilità ribadita dal Governo ieri in questa Aula al nostro emendamento che, nel merito, chiedeva di aumentare le risorse finanziare a favore di Polizia, Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Guardia di finanza e Vigili del fuoco. altresì incomprensibile e inaccettabile il rifiuto ad applicare al personale delle forze di polizia e delle Forze armate la normativa sull'equo indennizzo in caso di infortuni ed incidenti sul lavoro secondo quanto previsto dalle leggi generali dello Stato a tutela dei lavoratori. Come Partito Democratico abbiamo già detto di ritenere fondamentale che il Parlamento lanci al Paese un segnale chiaro e netto di contrasto e di lotta alla criminalità di stampo sessuale, particolarmente contro quella perpetrata ai danni di minori e delle persone più deboli. Ma il Parlamento deve compiere ulteriori passi in avanti

in particolare, sulla tutela delle persone deboli e vulnerabili, sulla formazione culturale di giovani e ragazzi, sulla istituzione di servizi sociali e di sostegno anche psicologico appropriati, sulla creazione di programmi di prevenzione, di diagnosi e di intervento a favore delle vittime, sulla formazione specifica di squadre della Polizia giudiziaria in un'ottica di prevenzione, sui protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (Comuni, Province, aziende sanitarie, uffici scolastici, forze di polizia)

di lottare contro la violenza sessuale e a tutela dei minori e dei più deboli. È per questo che il nostro Gruppo voterà responsabilmente a favore chiedendo, fin d'ora, a Governo e maggioranza che l'opera intrapresa venga proseguita, perché è finito il momento della propaganda e degli *spot*: è il momento di norme concrete e di merito, che noi continueremo a proporre e a sostenere.

votare insieme al Gruppo e contro questo provvedimento non tanto e non solo per il metodo, cioè l'adozione di un decreto‑legge che impone al Parlamento di approvare un testo

un provvedimento che mostra i muscoli, che fa la faccia feroce e che quindi prevede maggiori pene (ergastolo, carcerazione preventiva obbligatoria), mentre in Italia ogni anno 140.000 processi cadono in prescrizione.

si realizza la violenza più grave (quella fisica e quella psicologica) contro le donne, passa invece indenne, diventa una sorta di zona franca tutelata di fronte alla violenza contro le donne vi sia bisogno innanzitutto di iniziative culturali, di rivoluzionare una società maschilista e paternalista. Non è certo con questa legge che le violenze contro le donne

che caratterizza la presenza radicale al Senato è già entrata la senatrice Poretti. Anch'io annuncio il mio voto contrario con rammarico, proprio perché non è la prima volta che su temi relativi alla giustizia dobbiamo votare in dissenso dal Gruppo del Partito Democratico, pur condividendo la stragrande maggioranza degli emendamenti proposti, a a differenza di altri Gruppi, come l'Italia dei Valori, che dicono di essere l'unica opposizione ma neanche quello fanno, per essere sempre e solo d'accordo - magari la notte piuttosto che il giorno - con il Governo Berlusconi. L'Italia è un delinquente abituale per l'amministrazione della giustizia davanti alla Corte dei diritti umani di Strasburgo: ogni giorno c'è una sentenza di condanna per il modo in cui i diritti civili degli italiani sono violati dal nostro sistema giudiziario. questo decreto non aveva niente della necessità, niente dell'urgenza e va ad aggravare una situazione in cui, piuttosto che inasprire le pene, bisognerebbe prendere in considerazione, come è stato fatto nella legislatura scorsa, non tanto o non solo un indulto, ma addirittura un'amnistia per concedere ai magistrati, ai giudici e a 10 milioni di italiani di poter finalmente vivere appieno

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, questo decreto, che la Camera ha in parte modificato e sulla conversione del quale il Popolo della Libertà in Senato esprimerà un convinto ed unanime voto favorevole, è stato oggetto nei giorni scorsi di tante e varie critiche, di interpretazioni e, consentitemi, gratuite ed esagerate esegesi. Prima di soffermarmi allora su ciò che queste norme realmente sono e sul loro perché, ritengo opportuno argomentare ciò che il provvedimento non è mai stato, se non nella mente e nella bocca di chi - in verità in maniera sempre più isolata - esprime demagogiche ed insostenibili, quanto fantasiose, valutazioni. Questo provvedimento non ha mai espresso alcun giudizio sull'immigrazione in quanto tale: siamo ben coscienti che i grandi fenomeni migratori non possono essere fermati. Nessuno è mai riuscito a fermarli. Nessuno - aggiungo io - ha il diritto di fermarli. Sono i vasi comunicanti della storia, che creano - ma solo col tempo - integrazione e sintesi tra i popoli. Non è necessario invocare un principio di solidarietà ma basta rifarsi alla storia italiana, fatta di immigrazione, di emigrazione, di conquiste e, a volte, di indimenticati soprusi subiti. abbiamo sviluppato una grande capacità di sintesi: da una parte l'orgoglio di essere italiani e dall'altro la straordinaria capacità di accoglienza e di rispetto dell'altrui dignità. Se è vero che i fenomeni migratori non possono essere fermati, tutti noi, viceversa, abbiamo un grande e difficile compito: quello di governarli, di mitigarne l'impatto, di consentirne la decantazione e di attutirne la iniziale devastante difficoltà e l'emergenza che ne consegue. È ciò che 1'Italia sta vivendo: qualcuno abbia il coraggio di negare in quest'Aula che siamo oggi in stato di emergenza, nel momento in cui si aprono continuamente nuovi fronti senza che alcuno si affievolisca. Questo provvedimento, colleghi, non ha mai scritto, nemmeno nella sua versione originaria, l'equazione immigrazione uguale delinquenza, ma piuttosto ha posto in termini concreti misure determinanti per la dignità dell'immigrato. Qualcuno pensa forse che si possa riconoscere a qualsiasi di noi l'identità di appartenente ad una comunità, etnica, culturale e sociale senza prioritariamente aver acquisito una identità individuale? Vi chiedo, colleghi, se può esistere dignità senza identità. Crediamo di no. Questo è un obiettivo primario. L'identità di ciascuno di noi è la garanzia della nostra stessa libertà, della sicurezza di tutti, del vivere civile. Nessun accanimento contro nessuno, quindi: questo principio di collaborazione nell'accertamento dell'identità da parte dell'immigrato e la possibilità di una proroga dei termini di permanenza nei CIE, come più volte il sottosegretario Mantovano ha spiegato, sono contenuti nella direttiva comunitaria 2008/115/CE e troveranno comunque applicazione in un altro provvedimento che si rende a questo punto necessario e ineludibile, come previsto da un ordine del giorno votato ieri in quest'Aula. D'altro canto, colleghi, l'aver espunto l'articolo 5 e parte dell'articolo 6 ci consente di varare oggi un provvedimento con un voto sostanzialmente unanime. Questo è un fatto importante perché, secondo me, dà sicurezza al cittadino. Il contenuto centrale e innovativo di questo decreto - e di questo ringraziamo il ministro Carfagna - è l'introduzione nel codice penale del reato di atti persecutori, di *stalking* *to stalk*, «fare la posta»), e l'inasprimento di alcune misure di contrasto alle violenze sessuali, in special modo contro le donne e i soggetti deboli. Vi confesso, però, che mi pesa molto pensare e definire la donna un soggetto debole: considero questa una vulnerabilità non ontologica ma emergenziale, in quanto generata da un vero allarme sociale. Tutti i reati, come i colleghi magistrati e avvocati ben sanno, hanno un andamento di curva sinusoidale: aumentano e diminuiscono nei diversi periodi. Le violenze sulle donne hanno un andamento crescente ormai da 15 anni, con una lieve flessione nell'ultimo anno. Ed anche gli oltre 230 casi di *stalking* denunciati dal momento dell'emanazione del decreto parlano di una realtà sommersa che stenta ad appalesarsi, ma che vuole esplodere, e di un nuovo, opprimente, pericoloso, grave disagio della donna nella società italiana. Ci sembra molto poco, se pensiamo che in questi giorni le donne afgane sono scese in piazza contro una legge che consente lo stupro in famiglia e per di più circoscrive l'efficacia di questa norma ad una sola etnia del Paese. La violenza di genere è una violazione dei diritti umani, anche se - lo dobbiamo ricordare - in Italia solo dal 1996 la violenza è reato contro la persona e non contro la morale. Norme più rigide di contrasto alla violenza sulle donne e sui minori e agli atti persecutori introdotti dal decreto erano quindi indispensabili, e non perché, come anche poco fa molti hanno detto, i *media* hanno voluto alterare, amplificandola, la percezione della collettività sulla gravità del fenomeno. Se anche ciò fosse vero, il cittadino avrebbe comunque il diritto di poter contare su serie e rassicuranti misure di contrasto. In realtà, queste si sono rese necessarie ed anche urgenti, soprattutto perché l'impunità di tali odiosi reati, agevolata da una percentuale di non denuncia che va dal 93 al 96 per cento dei casi, lascia di fatto in circolazione soggetti che dimostrano condotte pericolosamente recidivanti proprio ai danni dei soggetti più deboli. *PdL)*. Di qui, colleghi, l'opportuna scelta del Governo di intervenire con decreto (e di questo non dobbiamo sentirci offesi, senatore Li Gotti), capitalizzando il lavoro già svolto in parte dalla Camera e in parte dal Senato.

Non si può negare che il contatto con culture molto diverse dalla nostra, in cui la soglia di attenzione ai diritti delle donne e dei minori è molto bassa (ed in taluni casi è veramente molto bassa), aumenta il rischio; ma la maggior parte delle violenze, degli abusi sessuali e degli atti persecutori ora definiti dal nuovo articolo 612-*bis* del codice penale sono commessi in famiglia e da italiani, rivelando sacche impensate di frustrazione, disagio e nuove disperate solitudini. Questo è veramente il nodo della questione: mentre introduciamo rimedi, dovremmo insieme riuscire a comprendere la causa della malattia di una società sempre più violenta, insoddisfatta, disordinata e recalcitrante alle regole. Ho sentito che molti, in questi giorni, hanno voluto scomodare Beccaria per argomentare pene più miti ma certe, altri ancora hanno voluto ribadire la necessità del rapido svolgimento del processo. A tale proposito, vorrei ringraziare il ministro Alfano per la tempestività e l'intransigenza ancora una volta dimostrate

In ogni caso, la coscienza di un legislatore deve soffermarsi sempre anche sul perché certi fenomeni esplodono ed io so che tutti noi lo stiamo facendo, anche se le risposte che le nostre impostazioni culturali, ideologiche e politiche ci danno sono a volte coincidenti, più spesso diametralmente opposte. Penso comunque che la sicurezza del cittadino e la vivibilità delle città per le donne, i bambini e gli anziani, i cosiddetti soggetti deboli, passi anche attraverso la buona amministrazione della città e l'attenzione dovuta alla sicurezza: non solo videosorveglianza, come prevede il decreto, ma una nuova concezione degli spazi (specialmente quelli dedicati ai bambini), delle distanze e degli orari. Intanto, è non di poco conto il fatto che, grazie a queste norme, si applica la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso in occasione del delitto di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza di gruppo. È obbligatoria la custodia cautelare in carcere, quando parliamo di questi reati. Colleghi radicali, anche noi abbiamo molto riflettuto su questa norma; abbiamo paura che si instauri un automatismo, ma è ovvio che il tutto è basato su un principio di precauzione che scaturisce dall'allarme sociale. Ci rimettiamo alla prudenza del giudice nella valutazione dei gravi indizi. Inoltre, i benefici e le misure alternative sono concessi ai condannati per atti persecutori sulla base dell'osservazione scientifica della personalità condotta almeno per un anno. Le vittime dei reati legati alla sfera della violenza sessuale hanno il gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. E vorrei dire a chi ieri ha affermato il contrario che non si può pensare di dare il gratuito patrocinio in base alla denuncia dei redditi di una persona, e che lo si deve fare in base alla gravità del reato. Volete forse dirmi che

Un altro fatto importante che voglio ricordare è che si estendono alle vittime di atti persecutori le misure di protezione nell'assunzione delle prove. Due settimane fa lo abbiamo previsto per le vittime dell'usura; a maggior ragione era giusto prevederlo per questo tipo di reati. Nella discussione che in Commissione giustizia del Senato si era già sviluppata sui disegni di legge sullo *stalking* alcune perplessità si erano manifestate in ordine alla complessità dell'accertamento del reato da parte del giudice e sulla inequivocabilità della sua definizione. Appare di non facile valutazione il "perdurante e grave stato di ansia o di paura" o il "fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto"; lo stesso vale per la linea di demarcazione tra il tentativo e l'effettiva consumazione del reato. E sull'ammonimento da parte del questore si potrebbe aprire certamente un contenzioso amministrativo che sicuramente non aiuterebbe psicologicamente la vittima e l'effettivo, quanto tempestivo, perseguimento del colpevole. Ho voluto ricordare, seppur sommariamente, queste norme per significare in quale delicata sfera dell'intimità, sia della vittima che del reo, si inserisce l'accertamento. E se si allungasse il processo, certo, si rischierebbe di danneggiare ancor più la vittima e di rinvigorire nei malsani propositi e comportamenti il delinquente. Dobbiamo tener presente che chi commette atti persecutori è un soggetto psicologicamente instabile, frustrato, vendicativo, se non addirittura malato. E poiché molto spesso l'autore di atti persecutori e di violenze è un familiare, in queste circostanze si determina comunque, anche per la vittima, la necessità di rimuovere e cancellare pezzi della propria esistenza, delle proprie esperienze, delle proprie abitudini. Ci sono comunque altre frontiere da esplorare, in questo campo. Con alcune colleghe senatrici ci siamo chieste, forse più da donne che da parlamentari, se uno stupro ad opera di uno sconosciuto o una violenza incestuosa o da parte di una persona che si è amata configurino realmente lo stesso reato e se possano imprimere in una donna o in un minore la stessa indelebile sofferenza psichica e fisica. Talvolta la violenza fisica è un mezzo per fare violenza psichica e talvolta la frustrazione psichica è solo una reazione ad una violenza fisica. Questo deve essere valutato. Ci siamo anche chieste, per lo *stalking*, quali saranno le reali difficoltà di applicazione di una norma definita genericamente

da consolidare. E poi ci siamo chieste se non sia il caso di introdurre il reato di *gaslighting*, cioè di *mobbing* familiare, che è insieme concausa ed effetto della deflagrazione dell'istituto della famiglia. Oggi con questo voto voto consegniamo un risultato importante a tutti gli italiani, in particolare alle donne italiane e - lo sottolineo - a quelle non italiane in Italia. Però, cari rappresentanti del Governo, vogliamo confermare che non riteniamo esaurito il nostro impegno di legislatori su questi temi e, soprattutto, quello di percettori del disagio sociale e della domanda crescente di sicurezza, di giustizia e di tutela dei soggetti più deboli. Per questo continueremo a confrontarci con un occhio alla strada e l'altro alle aule dei tribunali. Concludo Concludo menzionando alcuni luoghi per evocare con drammatica potenza tragedie profonde che hanno scosso tutti noi: Roma, Parco della Caffarella, stazione di Tor di Quinto, Fiera di Roma; Milano, Stazione centrale, via Selvanesco; Caserta, Piedimonte Matese.

e tempestività. Da quel momento, però, per loro inizia il diritto a dimenticare, mentre per noi, onorevoli colleghi, è ancora più forte il dovere di ricordare.

e nel rafforzamento delle forze dell'ordine il suo punto di forza: credo che questa sia una delle migliori e possibili risposte all'aumento della criminalità. Al riguardo, si evidenzia chiaramente e in maniera inconfutabile tutto l'impegno del Ministero dell'interno e del nostro ministro Maroni, che è passato attraverso uno stanziamento di oltre 100 milioni di euro, oltre a quelli che già aveva finanziato lo scorso anno. Noi della Lega Nord, in verità, ne volevamo molti di più, avevamo previsto 150 milioni di euro, però alla Camera qualcuno ha pensato bene di stralciare questo provvedimento.

prima erano previste al massimo 24 ore, oggi siamo arrivati a 7 giorni e anche oltre in casi eccezionali, e questo è stato molto, ma molto apprezzato da parte delle forze dell'ordine.

per facilitare la sicurezza nel nostro territorio e contrastare la criminalità. Avevamo chiesto che i tempi di permanenza dei clandestini all'interno dei centri di identificazione ed il loro riconoscimento, la loro identificazione, capire chi sono queste persone, cosa fanno, da dove vengono, cosa vogliono, quali siano le loro intenzioni. Chiedevamo che tali tempi di permanenza fossero di almeno sei mesi, però questo da parte di qualcuno non è stato accolto molto bene. L'opposizione, la sinistra - ma non solo la sinistra, credo anche qualche franco tiratore, o, come qualcuno ha detto, qualche "franco traditore"

hanno preferito votare il cosiddetto emendamento Franceschini, che prevede la liberazione immediata di oltre 1.400 clandestini, clandestini, ma ciò è niente, perché questi 1.400 clandestini facilmente si confonderanno con l'oltre un milione di clandestini già presenti nel nostro territorio. E forse, se qualcuno ancora non l'ha capito, noi i clandestini nel nostro territorio non li vogliamo: vogliamo che queste persone se ne ritornino subito a casa loro.

dei senatori Casson e D'Alia, che magari sono anche bravi a fare il loro mestiere di senatori, ma sulla sicurezza, secondo me, hanno qualcosa da imparare.

contrastano il reato di abigeato in Sardegna. In quel caso va assolutamente tutto bene, se poi questa forma di controllo del territorio viene mutuata da qualche altra parte non va più bene.

del territorio. Vi assicuro che io sono uno tra questi, lo sto facendo da diversi anni e continuerò a farlo perché credo in questa forma di controllo del territorio. La Lega Nord, comunque, continua sicuramente perché apprezziamo la volontà del Governo e degli alleati anche di maggioranza - è giusto riconoscerlo - che hanno condiviso i i nostri ordini del giorno, sia quelli sui centri di identificazione ed espulsione immediata sia quelli sulle associazioni di volontariato; ringraziamo per averli per averli recepiti. La Lega Nord continua e continuerà con grande senso di responsabilità a difendere come sempre la sicurezza della sua gente. Una Lega come sempre determinata, ferma sulle proprie posizioni (non molliamo sicuramente),

finestra"). Onorevoli colleghi, accogliamo oggi con particolare affetto e vicinanza gli studenti della scuola media «Sabin» di Capistrello, in Provincia dell'Aquila. Che la loro presenza in Senato rappresenti per tutti noi quella speranza di rinascita che dobbiamo alimentare con costanza, forza e impegno istituzionale. Grazie di essere qui oggi con noi ad assistere ai nostri lavori.

Presidente, ho ascoltato con attenzione il dibattito e, tra gli altri, anche l'intervento del mio collega Li Gotti che mi ha fatto capire alcune cose. Ho sentito l'ultimo intervento dove si rivendica con una certa *verve*

per la violenza carnale, ma in realtà lo rende facoltativo o sfuma l'analisi sui reati che riguardano i minori. Ne ricavo, di fronte all'indifferenza dell'Assemblea, della maggioranza e del Governo nei confronti di questo punto, che di fatto, nel silenzio, nell'indifferenza, e forse nella trascuratezza, sta passando una misura che non punisce la pedofilia. Mi chiedo se sia possibile ricevere una risposta in merito e, in ogni caso, per questo motivo non posso votare favorevolmente, quindi mi astengo.

soltanto oggi, 17 giorni dopo il terremoto che ha colpito la Regione Abruzzo in generale e la Provincia dell'Aquila in particolare. Non posso non sottolineare l'immensa costernazione che questa tragedia ha provocato nel mondo, tra i circa 1.300.000 abruzzesi d'origine ed emigrati, tra i 5 milioni di italiani all'estero e tra le comunità dei Paesi dove noi viviamo. La lontananza, le informazioni obbligatoriamente frammentate, il profondo affetto che coltiviamo per la nostra terra d'origine, per le nostre radici, sono tutti fattori che amplificano lo sconforto per il dramma che ha colpito tutta la comunità nazionale. Siamo però orgogliosi dell'esempio di solidarietà nazionale espressa da migliaia di volontari di tutta Italia e dell'efficienza dimostrata dalle istituzioni, dalla Protezione civile, dai Vigili del fuoco e da tutte le forze dell'ordine. A loro tutti va il più sentito e affettuoso ringraziamento da parte degli italiani all'estero. In tutto il mondo sono in corso migliaia di iniziative di raccolta fondi da destinare alla ricostruzione dell'Abruzzo, la terra dove peraltro io sono nato. Al fine di garantire la massima efficienza e la trasparenza nell'utilizzo degli aiuti provenienti dagli italiani all'estero, per i quali fanno da tramite le innumerevoli associazioni, le organizzazioni, i COMITES e il CGIE, ho chiesto alla presidente della Provincia dell'Aquila, Stefania Pezzopane, al sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, e al presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, di istituire nei prossimi giorni una commissione da porre a totale disposizione dei responsabili della raccolta dei fondi proveniente dagli italiani all'estero al fine di: non disperdere le risorse; effettuare interventi non sporadici, ma organici a un piano generale di ricostruzione; assicurare i donatori del buon esito del loro gesto di solidarietà; mettere i comitati e i responsabili delle risorse raccolte nella condizione di decidere liberamente cosa fare per gestire direttamente direttamente l'operazione; proteggere il più possibile il contributo degli italiani all'estero da ogni sorta di strumentalizzazione. La presidente Pezzopane ha già comunicato il suo accordo e non vi sono dubbi

Anche questa volta daremo il nostro contributo alla rinascita della Provincia dell'Aquila, dell'Abruzzo e continueremo la nostra paziente e infaticabile partecipazione allo sviluppo dell'Italia. Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la mozione presentata con 105 firme di senatrici e senatori del Partito Democratico e del Gruppo Misto punta a risolvere alcuni problemi drammatici per gli italiani all'estero, aggravati dalla legge finanziaria approvata l'anno scorso. I tagli indiscriminati ai vari Ministeri hanno creato una situazione di emergenza su tutti i capitoli del Ministero degli affari esteri di pertinenza della direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie. Per brevità di tempo ne ricordo solo i principali: un taglio di 17.700.000 euro per l'assistenza ai nostri emigrati di prima generazione, che penalizza soprattutto coloro che, nati in Italia, oggi risiedono in America Latina in condizioni di reale povertà e privi di assistenza sanitaria, sanitaria, aspettando la fine della loro vita; un taglio di 19.500.000 euro per i corsi di diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo. Quest'ultimo taglio mette a rischio un':incredibile realtà la prospettiva che alla fine di questo anno scolastico più di mezzo milione di figli di italiani all'estero non abbiano non abbiano più l'opportunità di frequentare i corsi di lingua e cultura italiana. Se non c'è la lingua, non ci sono più rapporti. Tagliare la lingua a una comunità vuol dire recidere le radici, i legami affettivi, culturali, politici ed economici, nonché impoverire l'identità delle nuove generazioni. Complessivamente sono stati inflitti tagli per oltre 41.800.000 euro e sono previste ulteriori riduzioni per gli anni 2010-2011. Se non si rimedia tempestivamente a questa situazione vorrà dire di fatto che l'Italia rinuncia ad avere rapporti con i suoi cittadini residenti Potersi avvalere dell'enorme risorsa rappresentata dall'impiego di alcune decine di milioni di euro per gli italiani all'estero è sicuramente l'investimento più redditizio al mondo, tenuto conto che, quantificato che, quantificato in moneta sonante, il contributo che gli italiani all'estero apportano all'economia italiana è stimabile nell'ordine di miliardi di euro. Porto un solo esempio: la sola Cassa di

che sono soldi prodotti all'estero e versati in casse estere ed investiti e consumati nell'economia italiana. A questo vanno aggiunti - cosa non quantificabile

I prodotti italiani si trovano in tutto il mondo non perché le aziende italiane hanno sviluppato un *marketing* geniale, ma solo perché milioni di italiani hanno richiamato questi prodotti ed oggi hanno aperto mercati di valore inestimabile. Nella mozione, che - me ne rendo conto, colleghi - è lunga e che mi auguro abbiate comunque letto, ho tentato di dare più informazioni possibili. Altri Paesi, come la Francia e la Germania, per esempio, in proporzione ai loro residenti all'estero, investono fino a dieci volte più dell'Italia. Siamo coscienti che urge una riforma generale della presenza italiana nel mondo. La madre di tutte le riforme, però, è quella del Ministero degli affari esteri, e bisogna avere il coraggio politico di affrontare questa riforma. Oggi anche gli organi di rappresentanza, gli istituti di cultura, la gestione dei corsi di lingua e cultura italiana, le scuole italiane, gli istituti di assistenza devono essere riformati, ne siamo coscienti. Non bisogna però distruggere tutto, perché tutto ciò che si distrugge oggi per superficialità e sottovalutazione non si potrà mai più ricostruire. Sono già stati licenziati centinaia e centinaia di insegnanti di lingua e cultura italiana nel mondo. Bisogna oggi, ora, dare una risposta certa da portare da portare avanti per i prossimi tre anni, il tempo necessario per fare le riforme che sopra ricordavo. Signora Presidente, questa mozione non è e non vuole essere una mozione contro qualcuno o qualcosa, ma vuole essere la risposta dell'Italia, del Senato della Repubblica italiana ai suoi cittadini nel mondo alla banale domanda: l''Italia vuole mantenere, sviluppare, rafforzare i suoi rapporti con gli italiani che vivono nel mondo? Sì o no? Di questo si tratta. Se la risposta fosse no, gli italiani all'estero ne prenderanno atto e andranno avanti nel loro percorso di integrazione nei Paesi di residenza, sperando che invece non si traduca poi in una sterile assimilazione. Se la risposta, come fortemente auspico, fosse invece sì, allora l'Italia dovrà ripristinare realmente e immediatamente i fondi per i capitoli del MAE di pertinenza della Direzione generale per gli italiani all'estero per gli anni 2009, 2010 e 2011, intraprendendo anche la strada delle riforme, al fine di rendere operativo questo investimento. Non si può rispondere alle migliaia di italiani all'estero con un generico impegno da parte del Governo, perché gli italiani all'estero hanno sempre risposto e contribuito allo sviluppo del nostro Paese con fatti tangibili, con concrete rimesse economiche, con risorse vere; è legittimo da parte loro aspettarsi oggi una risposta certa nei tempi e chiara nella sua quantificazione. Questa domanda, ripeto, non la poniamo ad una opposizione, alla maggioranza o al Governo; la poniamo al Senato, ai senatori della Repubblica italiana; dubito che ci sia qui in Aula un senatore che non conosca la storia dell'emigrazione e che non sappia cosa ha rappresentato l'emigrazione per il nostro Paese. Questa è la domanda, care colleghe e cari colleghi, che pongo a voi in quanto senatore, al di sopra dei vostri schieramenti politici.

Colleghi, ricordo che alle ore 12 si svolgeranno le votazioni per le elezioni dei Consigli di Presidenza della Giustizia tributaria, della Giustizia amministrativa e della Corte dei conti.

la mozione a firma dell'Italia dei Valori, che reca oggetto la disciplina degli italiani all'estero, contiene una proposta coraggiosa, moderna e a mio avviso necessaria. indubbio che sia sempre più essenziale una riforma capace di incidere e portare efficienza nel panorama delle forme e degli istituti di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero. Il bisogno di razionalizzare la rappresentanza e privilegiare quelle forme di promozione e tutela degli interessi delle nostre comunità all'estero che funzionano davvero è sostenuto dalla più ampia pubblicistica, dai giuristi della materia e dai mezzi di informazione, che riportano quotidianamente sprechi ed inefficienze o, peggio ancora, sperperi a fini clientelari di soldi pubblici. Ma una riforma ce la chiedono anche i cittadini, e mi riferisco, tra le altre, alle due petizioni all'esame della Commissione affari esteri. Anche il nostro Parlamento, inoltre, ha sentito questo bisogno ed anche il Governo. Infatti, con il cosiddetto decreto milleproroghe, approvato al Senato l'11 febbraio scorso, la durata in carica del mandato di due dei principali organi rappresentativi degli italiani all'estero, il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), è stata prorogata per ulteriori cinque anni, rinviando il rinnovo elettorale, che era per legge previsto nel marzo 2009. Nella relazione illustrativa di questo atto il Governo afferma, fra le motivazioni, che il posponimento è dettato dal fatto che è già in corso una riflessione parlamentare sul riordino della materia e che quindi non avrebbe senso procedere alle elezioni se poi si pensa alla modifica o alla soppressione di questi organismi, in quanto i membri eletti non sarebbero più legittimati a rappresentare gli italiani all'estero e si sprecherebbero così risorse che in questo momento appaiono sempre più preziose. Permettetemi qui di affermare come l'atteggiamento del Governo sia contraddittorio, a volte schizofrenico, quando con il decreto milleproroghe valuta giustamente le esigenze di risparmio con quelle dell'esercizio del voto e poi, sul *referendum* e sull*'election* *day*, ignora le stesse giuste riflessioni fatte a febbraio scorso, cioè prima della tragedia in Abruzzo, a seguito della quale vi è ancora più urgenza e necessità di utilizzare al meglio i fondi

Dunque, accertata la necessità di provvedere ad una riforma della materia, bisogna domandarsi su quali direttrici si vuole operare. Si deve tendere, cioè, all'efficienza, tagliando laddove non serve e premiando quelle forme di rappresentanza che invece funzionano oppure la nostra azione deve indirizzarsi verso il mantenimento di una struttura farraginosa

che utilizzare al meglio le nostre risorse pubbliche sia un dovere che come legislatori abbiamo nei confronti dei contribuenti; un dovere che dovremmo sentire anche verso quei cittadini che vivono fuori dai confini italiani e partecipano alla nostra economia pubblica con rimesse e versamenti nelle casse pensionistiche estere, il cui impatto, per quanto si legge nella mozione Micheloni, arriva

sopprimere questo ente che, come avrò modo di illustrare in seguito, appare assolutamente pleonastico, stante le recenti modifiche istituzionali apportate alle forme di rappresentanze e considerate le mutazioni occorse al fenomeno dell'emigrazione.

che le funzioni assegnate al CGIE nel 1989 sono ormai state sussunte da altri organismi di rappresentanza è dettata dalla istituzione della circoscrizione Estero e dall'elezione dei rappresentanti parlamentari dei cittadini italiani residenti all'estero, operata dalla legge del 27 dicembre 2001, n. 459. Le legge attributiva del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero è, come si afferma nella mozione, la naturale manifestazione di quel principio costituzionale espresso dall'articolo 67 della nostra Costituzione (che recita: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»), in quanto individua nel parlamentare in genere - ed in quello eletto nella circoscrizione Estero in specie - il rappresentante *erga omnes* delle comunità delle comunità italiane radicate fuori dai nostri confini. Tale rappresentanza è la massima espressione di rappresentatività democratica di cui il nostro sistema si è dotato, eliminando una discrepanza ed una disparità di trattamento dei diritti dei nostri cittadini che si protraeva dalla nascita della Repubblica. Si tratta, oggi, di assegnare effettivamente agli eletti all'estero quei ruoli rappresentativi, con vantaggi indubbi per i nostri connazionali. In particolare, con la creazione della circoscrizione Estero, vengono assorbite tutte le funzioni di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero che, a a seguito della riforma elettorale, appaiono realizzate dal CGIE tramite poteri rappresentativi minori rispetto a quelli - assoluti - assegnati invece dalla Costituzione alla figura del parlamentare, attorno al quale proprio per tale suo mandato istituzionale e costituzionale - dovrà necessariamente ruotare la riforma legislativa da affrontare, consacrandolo come elemento fondamentale di raccordo tra le esigenze delle comunità italiane all'estero e le istituzioni centrali. Se poi andiamo a vedere le altre funzioni che la legge n. 368 del 1989 affida al CGIE, oltre a quelle testé illustrate e assorbite dal parlamentare, troviamo le competenze maggiormente finalizzate allo sviluppo delle potenzialità a livello locale delle comunità italiane nel mondo e delle loro risorse economiche, culturali e sociali. Tuttavia, analizzando il panorama degli organismi dettati alla tutela e promozione degli interessi italiani nel mondo, si osserva che le stesse esigenze locali possono essere portate avanti con maggiore incisività ed efficienza dall'altro organo rappresentativo presente, ossia i Comitati I COMITES, infatti, sono più vicini alla popolazione poiché sono composti da membri eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3.000 connazionali, e non eletti in seconda istanza come i membri del CGIE. L'attento esame del testo delle due leggi sui COMITES e sul CGIE mostra una sostanziale identità di compiti e di funzioni in capo ai due organismi, qualificati entrambi come «organo di rappresentanza degli italiani all'estero» (legge COMITES, articolo 2) ed «organo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero» (legge CGIE, Per quanto riguarda le funzioni specifiche che gli articoli 2 e seguenti della legge n. 368 del 1989 affidano al CGIE, si può asserire senza incertezze che al momento le stesse vengono efficientemente portate avanti dai COMITES. Questi ultimi, infatti, contribuiscono, attraverso studi e ricerche, ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale, civile della comunità di riferimento e intrattengono perciò rapporti di collaborazione con i sindacati e la stampa locale. I Comitati sono inoltre chiamati a cooperare con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti all'estero. all'estero. Si chiede che i COMITES siano potenziati, che le loro funzioni siano valorizzate, per farne ancora di più il perno gravitazionale, a livello locale, delle multiple istanze provenienti dalle comunità degli italiani. Si chiede, inoltre, di aumentare la trasparenza e la responsabilità nei confronti degli elettori, anche tramite una modifica alla legge ... *(Il microfono prego di concludere una relazione annuale che contenga l'evidenziazione delle maggiori problematiche sperimentate dalla comunità di riferimento, da allegare al rendiconto consuntivo e al bilancio preventivo.

Per quello che riguarda invece i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, nella mozione dell'Italia dei Valori si sottolinea la necessità di rendere più agevoli e sicure le procedure volte a consentire l'esercizio del voto ai cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la dotazione di una moderna strumentazione tecnologica che permetta un pieno funzionamento dell'AIRE. Cari colleghi, vedete dunque che molto si può fare e molto si deve fare per migliorare all'interno un sistema di rappresentanza degli italiani all'estero. Questo lo dirò

Signor Presidente, tutto quanto è stato detto si riferisce non a una presenza marginale degli italiani all'estero, ma ad una presenza che supera i sei milioni di persone fra quelli che sono all'estero e quelli che hanno un'origine italiana e si trovano ugualmente all'estero. Questi milioni di persone che costituiscono la nostra emigrazione stanno fortemente cambiando. L'emigrazione tradizionale, che che vedeva i nostri padri imbarcati sulle navi per andare a cercare fortuna al di là degli oceani e che ha, comunque, conservato anche oggi un forte attaccamento e un forte rispetto

Grazie,

promuovendo una possibile sinergia fra questi istituti, enti e associazioni che non devono disperdere la loro azione, ma la devono concentrare e valorizzare. È stato detto che il momento dell'economia mondiale è europea non favorisce questo sforzo dal punto di vista finanziario. Eppure, vi sono dei modi per accrescere le disponibilità finanziare per realizzare queste azioni. Non mi riferisco soltanto ai risparmi di spesa che pure,

proporzionato a quanto possiamo fare. Dietro a questi mezzi che noi dobbiamo trovare, tagliando le spese inutili, promuovendo una concentrazione delle nostre azioni e, soprattutto, cercando nuovi strumenti di intervento finanziario, dobbiamo fare in modo che che ci sia una presenza italiana supportata da un Paese moderno che oggi, fortunatamente, ha acquistato un prestigio e una posizione internazionale che non ha mai avuto. Sfruttiamo questa nostra attuale posizione per rendere anche un servizio a chi, tra i nostri connazionali, abita in altri Paesi. *(Applausi

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la mozione sugli italiani nel mondo, firmata da 105 senatori del Partito Democratico e del Gruppo Misto, posta all'attenzione di quest'Aula non è tanto un documento sulla composita natura, le esigenze e le aspettative dei nostri concittadini all'estero, quanto un'opportuna e doverosa presa di coscienza di un fatto fondamentale nella storia e nella democrazia del nostro Paese: e cioè che l'Italia non è circoscritta ai 301.317 chilometri di 61 milioni dei suoi residenti (immigrati, parte integrante della Nazione, inclusi), ma si estende ad un'altra dimensione reale, viva e operante oltre i suoi confini. Si estende all'altra Italia, a quell'Italia che è il risultato, in 149 anni di unità nazionale, di una diaspora attraverso i cinque continenti abitati, equivalente all'odierna popolazione residente sul territorio della penisola. Ben al di là della retorica, per qualche verso inevitabile e perdonabile in occasione di discussioni di questo genere, l'opportuna e doverosa presa di coscienza alla quale ho appena accennato si rende tale dalla constatazione che dentro e fuori dalle nostra aule parlamentari c'è ancora chi storce il naso al tardivo atto di giustizia del riconoscimento e dell'applicazione del diritto di voto politico attivo e passivo degli italiani all'estero. Non solo si mette in dubbio e nella peggiore luce possibile l'esercizio di un inalienabile diritto democratico e costituzionale degli italiani, dovunque risiedano nel mondo, con argomentazioni intrise o di ignoranza, o di malafede o di viete discriminanti ideologiche, ma anche si nega dal Governo, in particolare dall'attuale Governo, un insieme adeguato e vitale di risorse e strumenti di una vera politica per gli italiani all'estero, cioè di una politica di attenzione per una parte inscindibile ed altamente qualificata della stessa Nazione. Ed è appunto alla palese ingiustizia, perpetrata con i selvaggi tagli dell'ultima finanziaria (proiettata con una mostruosa blindatura sull'intero triennio 2009-2011) ai capitoli di spesa della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero per gli affari esteri, che con la mozione in oggetto, di cui è primo firmatario il senatore Micheloni, nella parte finale (e direi essenzialmente centrale) dell'elaborato, si chiede al Governo di porre il minimo rimedio, stanziando finanziamenti integrativi, pari a meno di 42 milioni di euro che, nonostante l'innegabile gravità del momento economico generale, rappresenta una modestissima, quasi insignificante, componente del bilancio complessivo dello Stato. Sarebbe persino troppo generoso considerare selvaggio l'ingiustificabile e punitivo taglio del 60 per cento al bilancio per gli italiani all'estero, passato dai 73 milioni di euro del 2008 ai 28 milioni di quest'anno, con le seguenti riduzioni: da 34 milioni a 14 milioni e mezzo di euro per i corsi di lingua italiana nel mondo (e dobbiamo sorbirci anche la dichiarazione del nostro Ministro degli affari sul rilancio mondiale di lingua e cultura italiane); da 3 milioni e mezzo a 996.000 euro per le attività culturali;

Che si tratti di economie non solo discriminatorie per una parte precisa dell'entità e identità nazionale, ma anche false e controproducenti per gli interessi nazionali generali, è facile dimostrarlo con le cifre alla mano, anche se impossibile nei limiti di tempo concessimi. La domanda cruciale che in sintesi pone la mozione è se sia giusto, ragionevole, considerare un peso, e non una risorsa, gli italiani all'estero. Lo si vada a chiedere alle 74 Camere di commercio italiane dell'Assocamerestero presenti in 48 Paesi, con 24.000 imprese associate, in massima parte costituite da operatori commerciali e industriali italiani residenti all'estero, che sono importatori e promotori di prodotti, tecnologie, attrezzature, componentistica industriale dell'Italia odierna. Lo si vada a chiedere agli analisti dell'*export* italiano di generi alimentari, abbigliamento, autovetture e *design*, in prima istanza e in misura preponderante utilizzato da italiani permanentemente residenti all'estero. Lo si vada a chiedere alle centinaia di migliaia di ricercatori, studiosi, tecnici, imprenditori, creativi italiani in tutti i settori di umana attività operanti nel mondo. Lo si vada a chiedere, ad esempio, agli italiani del Sudafrica, con i quali sono stato negli ultimi giorni, che con voce univoca, da Johannesburg a Città del Capo, a Durban, a Pretoria, ci tengono a chiarire di essere non una comunità di emigranti, ma una comunità di imprenditori. Lo si vada a chiedere, per fare l'esempio di un altro territorio della mia ripartizione elettorale, all'organizzazione del Forum dei parlamentari italo-australiani, i quali, sulla base della massiccia presenza italiana in Australia, sono stati l'elemento trainante per la creazione di un'esemplare democrazia multiculturale. Lo si vada a chiedere, ancora, ai milioni di nostri concittadini che, con la loro emigrazione e le loro rimesse, non solo contribuirono sostanziosamente alla rinascita economica di intere Regioni d'Italia nel secondo dopoguerra, ma che ancora oggi, come esplicato in un brano centrale illuminante della mozione, costituiscono, costituiscono, con versamenti di natura sia privatistica che pubblica, la fonte di un fiume aureo valutato in circa 5 miliardi di euro all'anno: tanto per sfatare una volta per tutte il mito degli italiani all'estero che non pagherebbero le tasse e che pertanto non avrebbero diritto neppure ad una rappresentanza elettiva. Per concludere, gli italiani nel mondo hanno dato e continuano a dare in misura ben più ampia di quanto non abbiano finora ricevuto e chiedono (chiedono, e di doveri, risorse per strumenti di ulteriore valorizzazione di questa magnifica realtà, semplici atti di giustizia e meritato riconoscimento.

onorevoli senatori, l'Assemblea del Senato affronta oggi la tematica degli interventi e degli strumenti a sostegno delle collettività italiane all'estero. Le mozioni parlamentari, presentate rispettivamente da senatori di maggioranza e di opposizione, segnalano con efficacia l'attenzione del nostro ramo del Parlamento sul punto, di grande importanza e attualità nello scenario politico, al di là del colore politico e dell'appartenenza partitica. Il mio ruolo di presidente del Comitato per le questioni degli italiani all'estero fa sì che io non possa esimermi dal sottolineare alcune problematiche che interessano le politiche per gli italiani residenti all'estero. Mi piace peraltro ricordare, preliminarmente, come anche sulla mozione parlamentare istitutiva dell'organismo che ho l'onore di presiedere, che recava le firme di senatori appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari, si sia registrato un consenso unanime, e ciò a dimostrazione di una continuità di interesse del Senato per l'approfondimento della conoscenza e per l'individuazione

l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero, nell'ambito della quale approfondire lo stato di attuazione delle normative e degli interventi, onde valutare modalità e tipologie di eventuali novelle e di più incisive strategie di disciplina e sostegno. Il Presidente ha già autorizzato lo svolgimento di detta procedura informativa, che sarà pertanto avviata al più presto. Vorrei anche richiamare il fatto che delegazioni del Comitato, composte in modo tale da rappresentare maggioranza e opposizione, hanno partecipato, negli scorsi mesi, ai lavori delle Commissioni continentali del Consiglio generale degli italiani all'estro (CGIE). In particolare, le delegazioni hanno preso parte alle riunioni della Commissione Europa a Costanza, Paesi anglofoni extraeuropei a Brisbane e America Latina a Buenos Aires. L'esperienza riportata dai senatori costituisce una preziosa visuale diretta sui sentimenti e sulle esigenze che vengono segnalate nell'ambito di quei Paesi in cui la presenza dei nostri concittadini è più radicata e consistente. Le problematiche che sono emerse con maggiore pregnanza riguardano, principalmente, la preoccupazione per la riduzione degli stanziamenti dedicati ai capitoli di bilancio per gli interventi per gli italiani nel mondo, per l'anno in corso e nella proiezione triennale della manovra di finanza pubblica. Tra i settori maggiormente toccati dalla diminuzione degli stanziamenti vi è quello del sostegno alla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero e quindi agli enti che gestiscono gli insegnamenti e agli istituti di cultura. Ulteriori problematiche sono quelle che si pongono in relazione all'assistenza ai nostri connazionali indigenti che vivono all'estero, nonché all'individuazione di apposite politiche destinate ai giovani italiani all'estero e alla terza età. Un'ultima tematica di stringente attualità è costituita dall'esigenza di procedere ad un riassetto della normativa in materia di rappresentanza politica dei nostri concittadini all'estero. Rispetto alle esigenze segnalate dalle nostre collettività nel mondo vorrei svolgere talune considerazioni di ordine generale, per poi soffermarmi su profili più specifici. Come ben evidenziato dalle premesse degli atti di sindacato ispettivo al nostro esame, i cittadini italiani emigrati all'estero hanno da sempre costituito un elemento di primaria importanza e di ricchezza per il nostro Paese. Vorrei segnalare che la mia Regione, la Sicilia, è una delle aree del Paese di più consistente provenienza dei flussi migratori. Quella siciliana, ad esempio, è la prima comunità per consistenza numerica in America Latina. Peraltro, i passi iniziali del fenomeno migratorio si riconnettono alla stringente necessità per gli emigrati italiani di procurarsi migliori condizioni di sussistenza e maggiori opportunità dal punto di vista lavorativo. A partire dalla ricostruzione susseguente al secondo conflitto mondiale, le rimesse provenienti dai migranti hanno consentito in molti casi la sopravvivenza dei nuclei familiari ancora residenti in Italia e hanno sempre contribuito in misura significativa al rilancio economico del Paese. Le successive generazioni hanno avuto l'opportunità di integrarsi nel tessuto economico e sociale dei Paesi di destinazione, ma sempre forte è rimasto il collegamento con l'Italia. Questa tipologia tradizionale di emigrazione è oggi affiancata da un certo numero di cittadini italiani, spesso di giovane età e qualificati dal punto di vista

per poi far rientro in Italia con un maggiore bagaglio di conoscenze ed esperienze. Anche da quest'ultimo punto di vista, peraltro, le ripercussioni per l'Italia derivanti dalla presenza di connazionali all'estero non possono che essere positive: i migranti di nuova generazione possono sostenere le prerogative economiche e commerciali dell'Italia e favorire la collocazione del Paese nello scenario internazionale. Si pone pertanto per l'Italia l'esigenza di valorizzare il legame con le collettività nel mondo e il Parlamento può rivestire un ruolo importante di indirizzo e di impulso nei confronti del Governo. Il riconoscimento del diritto di voto per le elezioni politiche è stato un primo, importantissimo passo. Peraltro, quale parlamentare eletto in Italia, sento nella mia carica l'eguale responsabilità di dedicare grande attenzione per le politiche per gli italiani nel mondo, in quanto fattore della politica nazionale nel suo complesso. Sottolineo inoltre che proprio la presenza dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero rende necessaria la riforma dell'attuale assetto di rappresentanza degli italiani all'estero, incentrato sui Comitati degli italiani all'estero e sul Consiglio generale degli italiani all'estero. Il tema risulta di stringente attualità ove si consideri che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 207 del 2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), per il rinnovo dei COMITES e del CGIE devono tenersi entro il 31 dicembre 2010, secondo le nuove modalità stabilite dalla riforma normativa. La Commissione esteri del Senato sta esaminando le proposte legislative in tale materia e il Comitato per le questioni degli italiani all'estero affiancherà con la propria attività conoscitiva e di approfondimento l'*iter* legislativo. Occorre conclusivamente notare, quindi, come la problematica delle politiche migratorie presenti aspetti tra loro strettamente interconnessi che vanno affrontati a livello onnicomprensivo. Il compito di sostenere tali politiche deve peraltro necessariamente misurarsi con il difficile contesto economico-finanziario in cui il Governo e il Parlamento si trovano ad operare. La crisi finanziaria ha imposto una linea di contenimento sul versante della spesa pubblica, che ha inciso proporzionalmente su tutti gli stanziamenti e quindi anche su quelli per la politica estera e per il sostegno alla missione di spesa dell'Italia in Europa e nel mondo. Pur alla luce di detto difficile contesto, il Parlamento può peraltro sottoporre all'attenzione del Governo l'esigenza di verificare l'attuabilità di interventi sulle tematiche di maggiore rilevanza per gli italiani all'estero. Mi riferisco ad una riorganizzazione del sistema alla

Tutto questo, Presidente, ci porta a considerare quanto importante sia oggi un'azione del Parlamento italiano rivolta ai nostri connazionali residenti all'estero.

«Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti»,

dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. Tale operazione avverrà a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento, sulla seguente lista compilata sulla base delle designazioni pervenute dai Gruppi: Avvocato Marco Baldassarri - Dottor Adolfo Cucinella. Ricordo che, in base alla citata disposizione di legge, i due candidati saranno proclamati eletti se la lista otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'Assemblea, cioè 162 voti. I senatori favorevoli alla lista proposta voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto,

e il dottor Adolfo Cucinella, ai quali rivolgo, a nome dell'Assemblea, i migliori auguri di buon lavoro. *(Generali applausi).* Passiamo ora alla votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa,

Tale votazione avverrà a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento, sulla seguente lista compilata sulla base delle designazioni pervenute dai Gruppi:

Procediamo ora alla votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, e dell'articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205. Tale votazione avverrà a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento, sulla seguente lista compilata sulla base delle designazioni pervenute dai Gruppi: Professor avvocato Beniamino Caravita di Toritto - Professor avvocato Angelo Pandolfo. Ricordo che, in base alla citata disposizione di legge, i due candidati saranno proclamati eletti

Proclamo eletti il professor avvocato l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto e il professor avvocato Angelo Pandolfo, ai quali rivolgo, a nome dell'Assemblea, i migliori auguri di buon lavoro.

Colleghi, possiamo procedere o dobbiamo sospendere la seduta?

intervengo con particolare interesse, visto che sono stata eletta nella Circoscrizione estero, in questa discussione sulla mozione d'iniziativa del senatore Micheloni, riguardante gli italiani nel mondo. Il nostro Gruppo parlamentare, avendo sottoscritto tale mozione, il cui tema è l'approfondimento della conoscenza delle diverse problematiche concernenti la crisi economica mondiale che coinvolge la collettività italiana all'estero, non potrà che votare a favore. Ho piacere, pertanto, di intervenire sullo stesso argomento che è stato al centro della riunione della Commissione continentale, tenutasi a Buenos Aires il 16 aprile scorso, e che oggi è in discussione in quest'Aula del Senato. Nel mese di febbraio la Commissione affari esteri si è riunita per svolgere un'audizione del senatore Mantica sulle problematiche degli italiani all'estero. Nel suo intervento è emersa una situazione alquanto difficile riguardo il futuro della nostra collettività. L'argomento fondamentale, attorno al quale ruota al quale ruota tutto il sistema degli italiani all'estero, è stato quello dei tagli alla rete diplomatico-consolare previsti sui capitoli di spesa relativi al triennio 2009-2011. Secondo quanto detto dal Sottosegretario, le riduzioni previste si aggirano intorno al 60 per cento dello stanziamento dello scorso anno. Sulla base delle considerazioni esposte nel corso dell'audizione, che senza dubbio mettono a rischio l'intera struttura politica riguardante gli italiani all'estero, ho affrontato nella Commissione continentale ed espongo anche qui alcuni punti che credo siano fondamentali per proseguire il lungo percorso intrapreso dalla nostra collettività all'estero, nella speranza di mantenere sempre vivo il senso d'appartenenza dei cittadini italiani di seconda e terza generazione. I temi di cui

I colleghi ritengono che questa discussione su una mozione di iniziativa di tutti i Gruppi sia importante oppure che non conti alcunché? Perché se non conta alcunché, è più dignitoso non fare queste discussioni,

Per quanto riguarda la promozione ed il sostegno della lingua italiana, a livello scolastico e culturale, se il Governo non interverrà prima di settembre per correggere i tagli, i corsi di lingua e cultura italiana scompariranno in tutto il mondo. Io credo che tutti questi tagli contribuiranno ad indebolire la figura degli italiani all'estero con conseguente riduzione anche nella diffusione del *made in Italy*, che toccherà tutti i settori, con evidenti ripercussioni negative sull'immagine e sull'economia del nostro Paese. Penso, inoltre, che sia opportuno rivolgere lo sguardo alle giovani alle giovani generazioni che rappresentano un punto di riferimento fondamentale, da non disperdere nel tempo, assicurando loro una partecipazione attiva all'interno dei COMITES.

un rinnovamento generazionale formato da giovani imprenditori, professionisti che rappresentano la realtà dell'emigrazione del ventunesimo Sono convinta che loro saranno in grado di confrontarsi con il cambiamento e contribuire, insieme a noi, alla costruzione di un Paese migliore.

Mi auguro che, con questa mozione, la collettività degli italiani all'estero, con l'aiuto di tutti noi parlamentari, dei membri dei COMITES, dei componenti del CGIE e del mondo giovanile, possa raggiungere un importante risultato per il futuro benessere di tutti i

un pensiero di tutti noi oggi dovrebbe essere rivolto a questi nostri connazionali che in un certo momento hanno lasciato l'Italia e che qui, in questa Aula in particolare - e non è la prima volta che lo dico - sono tutti

Signor Presidente, il senatore Micheloni ha già dettagliatamente illustrato i contenuti della mozione che lo vede quale primo sottoscrittore. un documento che il Gruppo del PD ha compattamente sottoscritto e che, nonostante siano trascorsi alcuni mesi dalla sua presentazione, mantiene inalterata, senza dubbio alcuno, la sua valenza politica; valenza politica dettata, in primo luogo, dagli effetti che si stanno determinando sulle politiche a sostegno dei cittadini italiani all'estero in conseguenza delle scelte adottate dalla maggioranza con la finanziaria del 2009. Si tratta dei cosiddetti tagli orizzontali nei vari capitoli di spesa che hanno toccato anche in modo considerevole questo settore. In secondo luogo, voglio osservare che, grazie alla presentazione di questo documento, il Senato è chiamato ad un confronto di merito su come il nostro Paese si propone di affrontare i problemi, le necessità e le aspettative di circa 4 milioni di cittadini italiani residenti all'estero. Da questo punto di vista risulta particolarmente significativo il fatto che l'Italia, con la scelta di ampliare ai nostri connazionali residenti fuori confine la rappresentanza parlamentare, ha mostrato una grande sensibilità politica ed istituzionale, al punto che altri Paesi stanno ora procedendo lungo quella direttrice, similmente appunto a quanto fatto da noi e dallo stesso Portogallo. e questo è il senso profondo della nostra iniziativa, si tratta di operare sul fronte delle politiche e delle conseguenti risorse da mettere a disposizione all'interno di un contesto sicuramente diverso anche dal più recente passato. un contesto che propone alla nostra attenzione il tema tutto politico di come il nostro Paese possa, anche a partire dalla grave crisi economica internazionale in atto, rispondere al meglio sul fronte di un'ancora più decisa e marcata valorizzazione di questi nostri connazionali, che sono protagonisti nei fatti della proiezione dell'Italia nel mondo e che contribuiscono direttamente alla diffusione della nostra lingua, della nostra cultura, delle nostre produzioni, con sicure e positive ripercussioni sull'immagine e sulla stessa economia del nostro Paese. Questo è lo spirito profondo che caratterizza il nostro posizionamento politico. Non ci muove la volontà di segnare una differenziazione aprioristica, si tratta al contrario di mettere in campo un comune volontà d'azione, che sappia, da un lato, rispondere alle necessità presenti e, dall'altro, delineare un quadro condiviso di azione tendente così a valorizzare l'interesse generale del nostro Paese. In questo quadro l'assunto da cui partire, e che credo sia condivisibile da tutti, è che i nostri cittadini migranti rappresentano una preziosa risorsa multiculturale per il Paese, un valore aggiunto che sarebbe deleterio non considerare nella costruzione di progetti e risposte ai temi ed agli interrogativi economici, culturali e sociali oggi presenti, in un contesto internazionale sempre più interconnesso, per usare un termine oggi molto in voga. Oltre alla necessaria e doverosa solidarietà nei confronti dei nostri concittadini che si trovano in condizioni di disagio, è del tutto evidente che oggi siamo chiamati ad affiancare gli interventi di natura assistenziale con azioni e conseguenti politiche che puntino a valorizzare ed a sostenere quelle esperienze, quelle professionalità e quelle conoscenze che caratterizzano oggi la presenza di moltissimi nostri connazionali nella vita sociale, economica ed anche politica dei vari Paesi di residenza. Allo stesso tempo, la politica a favore dei nostri migranti è oggi un campo d'azione di sicura importanza per la funzione del nostro Paese sul crinale della diffusione dei valori del dialogo, del rispetto e della tolleranza tra i popoli; i nostri emigranti, quindi, visti anche quali protagonisti nei vari Paesi di residenza di un'Italia che si propone come soggetto attivo e positivo nella costruzione di un nuovo ordine mondiale fondato sul multilateralismo e la cooperazione. riguardanti i nostri migranti crediamo non vadano quindi nella direzione di una completa assunzione del valore e dell'importanza di questo settore per il campo di azione complessivo del nostro Paese. Mettere così drasticamente in difficoltà l'opera e le attese di molti connazionali all'estero sul fronte dell'assistenza e della diffusione e conoscenza della nostra lingua, così come intaccare l'attività degli organi di rappresentanza, significa pregiudicare nei fatti l'intensa e fitta rete di rapporti che questi nostri concittadini hanno costruito nel tempo e, altresì, andare in netta controtendenza rispetto a quanto altri Paesi europei, come la Francia e la Germania, stanno facendo. A conclusione del mio intervento mi permetto quindi di auspicare che il Governo possa, già a partire da questa discussione, rivedere al più presto presto quei tagli e quelle decurtazioni, rimpinguando quei capitoli di spesa così tanto necessari alla vita ed all'attività associativa dei nostri connazionali.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, i nostri connazionali nel mondo costituiscono da sempre un fattore di grande importanza per la vita del Paese. Le ondate migratorie del secondo dopoguerra hanno visto un consistente numero di cittadini italiani recarsi all'estero, alla ricerca di condizioni di vita e di opportunità di lavoro migliori. Le rimesse degli emigranti alle famiglie rimaste in patria hanno apportato un significativo contributo alla ricostruzione del Paese e sostenuto l'economia nazionale. Le seconde e terze generazioni di cittadini italiani all'estero hanno rafforzato la consistenza delle comunità italiane nei Paesi di destinazione, principalmente collocate in Europa e in America Latina, e hanno vissuto problematiche legate al delicato equilibrio tra esigenze di integrazione nel contesto locale e di mantenimento del legame con la madrepatria. Rispetto alle caratterizzazioni dei primi flussi migratori, l'attuale connotazione degli spostamenti di cittadini italiani all'estero, soprattutto per quanto concerne le giovani generazioni, è decisamente diversa. Si tratta di persone che vedono nel trasferimento non necessariamente uno spostamento definitivo, ma anche solo transitorio, per esigenze di specializzazione negli studi o nel lavoro. La valorizzazione del legame con i nostri connazionali all'estero, ambasciatori italiani nel mondo, può ripercuotersi solo in senso positivo sul ritorno in termini di immagine e quindi di migliori opportunità sociali ed economiche per l'Italia nel contesto internazionale. Il nostro Paese ha quindi la responsabilità e l'esigenza di mantenere vivi e densi di contenuti i rapporti con le nostre comunità all'estero. Quanto alle modalità dell'impegno in questa direzione, spetta anche all'organo parlamentare assumere precipue iniziative a livello legislativo, oltre che predisporre linee di indirizzo per l'Esecutivo. L'introduzione della rappresentanza parlamentare delle collettività, mediante deputati e senatori eletti nella circoscrizione Estero, si muove in tale senso. E tuttavia questo segnale non esime anche gli altri componenti del Parlamento dal rivolgere la propria attenzione alle problematiche che interessano le comunità italiane nel mondo. Quale componente del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, istituito nella corrente legislatura mediante una mozione parlamentare sulla quale il Senato si è espresso in modo unanime, ho avuto modo di godere di un osservatorio privilegiato sul punto. Ho partecipato la scorsa settimana a Buenos Aires ai lavori della riunione della Commissione continentale per l'America Latina del Consiglio generale degli italiani all'estero e in tale sede ho avuto contezza delle tante problematiche e delle diverse esigenze che emergono nei contesti territoriali di maggiore presenza italiana. I rappresentanti dei nostri connazionali all'estero esprimono preoccupazione per la riduzione degli stanziamenti destinati dalla manovra di finanza pubblica per il corrente anno e per il prossimo triennio ai capitoli di bilancio per le politiche migratorie. Si è sostenuto che profili di particolare delicatezza sono costituiti dall'assistenza, anche sanitaria, dei cittadini italiani anziani ed indigenti,

ad una riduzione dell'insegnamento e delle iniziative di promozione culturale. Mi piace comunque ricordare che sono in corso di esame presso la Commissione affari esteri del Senato disegni di legge in materia di riforma dei sistemi di rappresentanza di cittadini italiani all'estero, al fine di renderli maggiormente efficienti e consentirne una migliore operatività. Sussistono infatti necessità di adeguamento di compiti e strutture dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)

La riforma deve essere definita con sollecitudine, stante il previsto rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE, disposto con l'articolo 10 del decreto-legge n. 207 del 2008, da tenersi entro il 31 dicembre 2010. da tenersi entro il 31 dicembre 2010. In conclusione, l'intera materia, a livello complessivo, delle politiche per gli italiani all'estero è in fase di rimeditazione. La struttura e l'articolazione degli organismi di rappresentanza politica dei nostri concittadini vanno adeguate all'introduzione del voto per le elezioni. Le risorse finanziarie per le politiche migratorie hanno risentito, peraltro, dell'impostazione generale della manovra finanziaria che ha operato una riduzione lineare dei capitoli di spesa destinati a ciascun Dicastero e, quindi, anche al Ministero degli affari esteri. Occorre ricordare che detti tagli sono stati previsti sul fronte della spesa pubblica a livello onnicomprensivo, a fronte di stringenti esigenze di bilancio, dolorose eppure inevitabili nella difficile congiuntura economica nazionale e internazionale. Ciò non toglie che in un'ottica realistica si possa procedere ad una riorganizzazione, in termini di razionalizzazione ed efficienza, della diffusione della lingua e cultura italiana all'estero, oltre che nel senso della continuità dell'assistenza ai nostri connazionali all'estero

Signor Presidente, mi consenta innanzitutto di rivolgere un ringraziamento a chi ha presentato le mozioni, a cominciare dal senatore Micheloni, perché è opportuno che questa Aula affronti un tema così importante come quello degli italiani nel mondo.

Poiché credo di avere molti difetti, ma che non mi manchi la chiarezza, vorrei anche rispondere in maniera molto precisa. Avendo un alto senso del rapporto morale e politico nei confronti degli italiani nel mondo, sono molto critico su alcune delle molte cose qui dette. Vorrei farmi intendere. Questo Paese - e lo diciamo con grande franchezza - ha sempre considerato la storia dell'emigrazione una storia di serie B e di cui vergognarsi. Credo che voler bene e pensare a quel ruolo dell'Italia nel mondo significa anche agire in questo Paese perché venga recuperata quella parte della storia che è intrinseca nella storia dell'unità nazionale; significa oggi discutere cosa vuol dire identità nazionale italiana in un mondo articolato, complesso, multilingue e multiculturale. Che cos'è oggi l'italiano nel mondo? Siete sicuri - è la mia domanda - che sia proprio l'italiano che fate emergere nel dibattito? Il senatore Randazzo nel suo intervento ci ha ricordato che nella sua esperienza in Sudafrica i sudafricani italiani gli hanno risposto di non essere emigranti, ma imprenditori.

Allora, forse, onestà intellettuale vorrebbe che cominciassimo almeno fra noi, per capirci e affrontare seriamente il problema, a dire che esistono comunità italiane nel mondo tra loro molto diverse, che il problema del Sud America e degli italiani in Sud America è un problema diverso da quello di coloro che vivono nei Paesi anglosassoni ed extraeuropei (dal Canada, all'Australia, al Sudafrica), così com'è diversa la comunità degli italiani all'estero in Europa, sui quali potremmo aprire un discorso su cosa significhi essere cittadini italiani nel momento in cui stiamo costruendo l'Unione europea e dovremmo sentirci innanzitutto cittadini europei. Lo dico perché questo mi pare il vero tema del dibattito, per rispondere alla domanda di Micheloni. L'aver organizzato la prima assemblea dei giovani italiani nel mondo a Roma

attenti, però, cercando di eliminare una parte di demagogia che a mio giudizio è quella che impedisce a tutti noi, Governo, maggioranza e minoranza, di affrontare con grande serenità il problema.

e chi mi conosce sa che anch'io sono in grande difficoltà, i tagli al bilancio per i corsi di lingua italiana. Però vorrei anche parlare delle scuole italiane nel mondo, con 1.200 insegnanti italiani che vanno all'estero e che costano una certa cifra; vorrei parlare degli accordi bilaterali sulla possibilità di inserimento della lingua italiana nelle scuole di altri Paesi; vorrei parlare di enti gestori. Se affrontiamo un problema, non cominciamo con Garibaldi e la storia patria. Parliamo dei problemi sul tappeto ed affrontiamoli. Ci sono delle riforme da fare. Ci sono molti interventi, non di tagli di spesa, ma di razionalizzazione della spesa secondo obiettivi di efficienza e di efficacia.

e che di questa quantità enorme 950.000 riguardano solo Argentina e Brasile, credo che discutere di cittadinanza non sia

italiana. Chi conosce quella realtà, anche chi va a Buenos Aires a parlare al CGIE, dovrebbe chiedersi il perché questa esigenza. Forse potrebbe rispondere al meglio

perché non si può invocare l'identità italiana per chi chiede il passaporto per risparmiare sulle tasse per entrare negli Stati Uniti. Anche di questo dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare di corsi di formazione

me - il Governo brasiliano ha inteso assumere un atteggiamento, che io definisco non certo amichevole, nei confronti dell'Italia sul caso Battisti e la grande comunità italiana, fatta da milioni di persone, non ha sentito il dovere di esprimere una parola sull'atteggiamento del Governo brasiliano nei confronti del loro Paese di origine. Non si può essere italiani solo quando si chiedono i soldi. Essere italiani significa partecipare alla vita di questa comunità nazionale, facendosi carico delle proprie responsabilità e anche godendo dei propri diritti, chiedendo, come pretendo, di reinserire nella propria storia nazionale la storia dell'emigrazione. Bisogna anche cominciare a ragionare seriamente. Lo dico con grande rispetto nei confronti dell'onorevole Tremaglia, che è ricordato

se ne apre una nuova. Non è un caso che questo Governo, e ringrazio in questo senso l'Italia dei Valori che ha presentato una mozione specifica al riguardo, e ringrazio coloro che hanno presentato

credo infatti sia serio pensare che esistono 5.500 associazioni di italiani nel mondo: evidentemente, qualche problema c'è. L'assessore all'emigrazione del Veneto ha recentemente dichiarato che provvederà a fare un censimento, perché, distribuendo 2,4 milioni di euro all'anno la Regione Veneto, non capisce più dove vadano a finire i suoi soldi.

una linea di indirizzo né un disegno di legge da imporre, ma vuole e pretende che questo dibattito nasca in Parlamento e siano le forze parlamentari ad indicare la modifica del sistema di rappresentanza; ovviamente farà la sua parte (di aiuto, di indirizzo e di consiglio) rispetto a coloro che lavoreranno, sostenendo che bisogna mantenere l'impegno del decreto milleproroghe e dimostrare che il Parlamento italiano è in grado

Mi consenta, però, il senatore Micheloni, che conosco, di dire che forse nel suo partito sarà meglio che ci si metta d'accordo, perché l'intervista

il rapporto tra i COMITES ed i consolati. A parte le insinuazioni che vi vengono fatte, occorre però stabilire che se i Comites sono autonomi rispetto ai consolati non si può chiedere alla Farnesina di intervenire nel loro scioglimento.

e mantenere, in quanto rappresentante dello Stato italiano sul territorio, una funzione perlomeno di controllo (perché credo che questo rientri nelle funzioni della Farnesina) e la più ampia autonomia (e dovremo discutere anche di questo in materia di

vi è sullo sfondo anche quello della cittadinanza, che cercheremo certamente di affrontare: mi pare però che molto più seriamente lo si debba affrontare dal punto di vista della cittadinanza italiana per coloro che oggi sono immigrati in Italia e quindi rivedere

anche dati veritieri. Cito un solo dato, che nessuno ha menzionato, visto che parliamo sempre male delle strutture del Governo italiano all'estero. Ricordo che gli istituti di cultura ricevono 22 milioni di euro dal Governo

vuol dire che la lingua e la cultura italiana si possono insegnare anche non gratuitamente. Infatti, non credo che 23.630.000 euro nel 2007 non siano un'importante cifra

ma vorrei che coloro che hanno presentato le mozioni capissero il senso della risposta, che va data, ovviamente, sulle cose scritte e non sulle intenzioni. Devo esprimere

che nella discussione parlamentare il Governo si augura che venga rivisto pesantemente il ruolo del CGIE, in gran parte superato dalla presenza dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero in questo Parlamento,

Mi auguravo che si potesse arrivare ad una mozione congiunta di maggioranza e opposizione, ma questo non toglie assolutamente nulla al valore di tutte le mozioni presentate. Per quanto riguarda la mozione della

Nel correggere l'impostazione del 2009 il Governo ritiene che la priorità assoluta vada data al problema dell'insegnamento della lingua italiana, anche per un motivo molto semplice che chi è addetto ai lavori conosce perfettamente. I tagli si misureranno non tanto su quello che è avvenuto, perché finora, da quanto ci risulta, si è riusciti a mantenere un livello quantitativo di corsi

caso, vorrei essere chiaro: le percezioni consolari sono quelle relative ai visti che il sistema diplomatico della rete consolare italiana dà nel mondo. Si tratta di una cifra importante; c'è una quota parte stabilita già assegnata al Ministero degli affari esteri, ma

chiudere questa partita destinando ai corsi di lingua italiana le risorse che dovessero pervenire. Concludo ringraziando comunque tutti gli intervenuti. Mi auguro che in Parlamento si possa

accanto ai parlamentari quando verrà richiesto il suo intervento. Credo che, se ripartiremo dalla riforma dei sistemi di rappresentanza e dall'allargamento della platea

alla domanda del senatore Micheloni - di valorizzare la presenza della comunità italiana nel mondo, nella costruzione di una più grande comunità nazionale, fatta da residenti in Italia e residenti all'estero, credo che in questa legislatura avremo compiuto un buon lavoro. apre una nuova finestra"). Prima di passare alla votazione delle mozioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione

il fenomeno dell'emigrazione dei cittadini italiani verso i paesi esteri ha subito, dal forte esodo dei primi anni del Novecento, trasformazioni rilevanti sia sotto il profilo della composizione sociale dei migranti,

su questo, ossia cerca di rispondere ai mutamenti accorsi al fenomeno dell'immigrazione sopra considerati rimodellando le modalità con le quali le nostre istituzioni si attivano al fine di presentare politicamente gli italiani residenti all'estero: valorizzare la nostra lingua, la nostra cultura, la nostra immagine nel mondo, incentivare l'economia del *made in Italy*, sostenere i mezzi di informazione locali all'estero e anche favorire il rientro delle conoscenze e delle esperienze realizzate dai cittadini italiani nella loro permanenza all'estero. La nostra mozione vuole appunto adottare un approccio per dialogare con gli espatriati; il livello locale di rappresentanza è dato dai COMITES mentre il livello globale,

La comunità italiana o di discendenza italiana che risiede all'estero rappresenta un pezzo importante della nostra storia. Oggi, l'apertura al mondo della nostra economia rappresenta la chiave del suo successo e di tutte le sue eccellenze. Gli italiani all'estero rappresentano da sempre, nei differenti continenti in cui si sono trovati, una vera comunità, solidale al suo interno, affezionata e nostalgica verso la propria terra. Si conserva l'uso della lingua e molto spesso all'italiano della scuola e della televisione si sostituisce nelle famiglie, magari quelle emigrate 30 o 40 anni fa, il dialetto locale; si conservano aneddoti e tradizioni, forse ancora più che in patria. Queste comunità sono molto spesso organizzate in vere e proprie forme di associazione che, nate come luoghi di ritrovo per sentirsi per sentirsi un po' più a casa, sono diventate negli anni reti di assistenza, di aiuto anche concreto fra i propri membri, di collegamento con le famiglie e con le comunità in Italia. Sono comunità molto strette e molto legate perché sono comunità che nascono dai territori omogenei, e non dalla legge di uno Stato: le comunità dei veneti, dei pugliesi o dei sardi non potranno mai essere soppiantate da forme istituzionali nazionali di nessun genere. A queste reti più vecchie, ma tuttora vivacissime, si stanno oggi affiancando nuove migrazioni, quelle dei giovani, che partono più come singoli che come gruppi rispetto al passato, certo per spinte economiche di tipo diverso, che sono meno organizzate ma meritano di essere supportate ed accompagnate perché rappresentano noi tutti nel mondo. Queste premesse brevi, e credo unanimemente condivisibili, chiariscono senza ombra di dubbio il grande valore e la considerazione che la Lega Nord attribuisce alla comunità dei concittadini residenti all'estero e alle politiche che possono incentivare e rafforzare il legame con il territorio nazionale e con i territori di origine. Ritengo tuttavia piuttosto riduttivo valutare la qualità delle nostre politiche verso i concittadini all'estero esclusivamente attraverso la quantificazione dei fondi assegnati. Quello che è stato fatto ad oggi dalla rete dei COMITES non ha dato i risultati sperati, indipendentemente dai fondi spesi.

il necessario sostegno a tutti i nostri connazionali residenti all'estero che versano in condizioni di difficoltà. Colgo l'occasione per ringraziare il sottosegretario Mantica perché ha preso a cuore questo problema delicato ed importantissimo.

che aveva il compito di progettare e sovrintendere alla realizzazione di una grande opera nazionale come il ponte sullo Stretto di Messina, a presentare tale opera ai cittadini italiani residenti in Nord America.

che avrebbero voluto siglare con la firma, mattone per mattone, di molte centinaia, se non migliaia di cittadini italiani, che si riconoscevano

corriamo il rischio di sottovalutare l'eccellenza, la forza e la determinazione dei nostri 60 milioni di connazionali di prima, seconda e terza generazione. Non è importante, signor Presidente, onorevoli colleghi, se la rappresentanza è affidata ai 4 milioni di cittadini che votano e hanno portato in Parlamento una ampia rappresentanza di deputati e senatori. A quei deputati e senatori è affidato oggi il compito di costruire un grande piano Marshall per il rapporto con l'Italia nel mondo, che non debba interessare solo quei quei cittadini iscritti all'Aire ma l'intera comunità di soggetti di origine italiana, che si ritrovano in una identità, in una bandiera, dinanzi alla quale perfino ancora piangono più di quanto a volte fanno i nostri connazionali residenti in Italia. La sottovalutazione riguarda l'impatto di sistema. Vedete, la mozione del senatore Micheloni e degli altri senatori del Partito Democratico parte da un'emergenza, quella del taglio dei fondi ad alcuni capitoli di spesa legati alla Direzione generale per gli italiani all'estero. Ma siamo di fronte ad una crisi terribile, che ha imposto sacrifici a tutta l'amministrazione dello Stato e pertanto era ipotizzabile che anche lì la scure della prudenza si sarebbe abbattuta su alcuni capitoli di spesa. Tuttavia, fa da contraltare a questo taglio la dichiarazione del ministro Tremonti: la crisi economica del nostro Paese sarà sostenuta con forza dalla determinazione dei nostri imprenditori italiani che lavorano nel mondo a rafforzare il proprio essere all'interno dei Paesi che ospitano il grosso delle nostre comunità italiane. Ne sono assolutamente convinto. Vedete: di fronte alla crisi che avvertiamo nel Paese la bilancia degli scambi delle nostre imprese, del *made in Italy*, non ha subìto ancora nei Paesi chiave delle contrazioni significative. Insieme agli imprenditori che da qui si muovono e che nei Paesi del mondo operano ci sono centinaia, migliaia di imprese di italiani all'estero che cooperano, sottoscrivano *joint venture*, contribuiscono ad espandere questo grande messaggio del *made in Italy*. Vi faccio qualche esempio: in Turchia, a nemmeno due ore di volo da qui, si stimano contratti per 17 miliardi in Russia, dove la comunità italiana non è molto estesa ma è costituita dall'eccellenza degli imprenditori, degli uomini del fare, si potrebbe arrivare a 30 miliardi di euro per rafforzare il già consistente bilancio del nostro fatturato d'impresa se solo investissimo sulla sede diplomatica e sui suoi addentellati consolari. Bisogna ragionare su quali investimenti fare all'estero. È vero che perdiamo dei fondi per per l'istruzione della lingua italiana, ma - l'ha detto il sottosegretario Mantica, che ringrazio per la chiarezza - si stanno moltiplicando le scuole dei Paesi ospitanti che insegnano l'italiano, e ciò per sollecitazione delle nostre strutture diplomatiche. Se in alcuni casi rafforzassimo invece che alcuni addentellati di spesa le sedi diplomatiche potremmo guadagnare più contrattazione commerciale, più turismo. Il rilascio dei visti non è solo un rilascio strumentale, come avviene in alcuni Paesi; ci potrebbe essere più turismo da Paesi chiave che guardano all'Italia come ad una meta importante e che stanno rafforzando la loro capacità di rilascio dei visti. Il dato della Turchia è di 400.000 visti rilasciati; lo stesso vale per la Russia. Se ci fossero più consolati ci sarebbe più traffico verso l'Italia. Si tratta di un'attività di sensibilizzazione che spesso riguarda, nei Paesi del Nord America e Sud America, nostri connazionali che vogliono gestire una sorta di operazione-ritorno verso questo Paese, nel quale

miliardi di euro in Italia, contribuendo alla rinascita economica del Paese. Ma dobbiamo aprire loro una strada. Ecco perché parlo di un piano Marshall rispetto alla percezione ed all'attività dei deputati e dei senatori presenti nel nostro Parlamento. Bisogna dargli una strada che superi i lacciuoli burocratici, che li indirizzi, per dire loro come, perché e quando si può investire dall'estero in Italia. Quelle risorse sarebbero significative per superare la nostra crisi economica interna. Faccio un esempio legato anche

raccoglierà le risorse per regalare alle popolazioni dell'Aquila cento appartamenti realizzati e finiti a propria cura, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile; un grande investimento, ma è una sola delle organizzazioni italoamericane di pregio ad intervenire. Immaginate quale sarà poi la prova di solidarietà degli italiani nel mondo nel loro complesso, che hanno fatto registrare una straordinaria presenza solidale a poche ore dai fatti dell'Abruzzo. Lo ha detto il presidente del Consiglio Berlusconi: rispetto a questa crisi economica nessuno resterà solo. E questo appello e questo impegno forte vale anche per gli italiani residenti all'estero: nessuno resterà solo, l'Italia continuerà a garantire, seppur seppur nel mutato quadro economico e finanziario, risorse per l'assistenza economica ed anche sanitaria ai nostri connazionali residenti all'estero che versano in condizioni di indigenza. In merito alla

A questo punto è naturale, come mi sembra di registrare da tutti gli interventi che sono stati svolti in tale discussione, immaginare una riduzione del numero dei COMITES, un adeguamento della CGIE alla mutata situazione ed un rafforzamento invece della rete diplomatica consolare sul territorio. Seguiremo ovviamente le istruzioni di rigore finanziario che il nostro Governo ha voluto darci. È una restrizione che ha portato risultati, inutile negarlo; è una restrizione che ci ha consentito di non subire danni al pari di altri Paesi europei. Ebbene, questa stagione di restrizioni è appartenuta anche al bilancio del Ministero degli affari esteri e della Direzione per gli italiani nel mondo, ma non sarà una stagione eterna: speriamo, con la presentazione di questa mozione, una mozione di speranza affidata al Governo, nella ripresa dei finanziamenti alle comunità italiane per l'insegnamento della lingua italiana e speriamo anche in una grande riforma dei meccanismi di rappresentanza...

Scusate, ci sono i senatori Segretari. Per favore, ritirate le tessere che non corrispondono

**Il Senato non approva.** I senatori Segretari hanno fatto un controllo e hanno ritirato le tessere

dedicati ai lavori della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, molto probabilmente - con un lavoro di regia che oggi avrebbe fatto vedere agli italiani chi hanno mandato in Parlamento con queste belle liste bloccate - in futuro una simile situazione non si ripeterebbe.